Signor Presidente, ringrazio gli interroganti. L'atto di sindacato ispettivo in oggetto solleva specifici quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità della casa circondariale di Brescia, Canton Mombello, con particolare riguardo alle carenze strutturali e organiche, al sovraffollamento, nonché relativamente al progetto di costruzione del nuovo penitenziario di Brescia, Verziano. Ancora una volta l'attenzione è giustamente rivolta al sistema carcerario, che da sempre rappresenta una priorità di questo Governo. L'emanazione del recente decreto "carcere sicuro", n. 92 del 2024, è la prova della risposta alla situazione cronica di emergenza degli istituti penitenziari e della volontà di creare un modello che assicuri certezza della pena, ma che non sia lesivo della dignità umana. Ricordo, tra le novità del decreto, la previsione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che avrà il compito di attuare in tempi rapidi il piano nazionale di interventi, sia per l'aumento dei posti detentivi sia per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di polizia penitenziaria. Venendo, nello specifico, all'istituto di Canton Mombello, dai contributi informativi resi dal DAP non sfugge che, malgrado gli interventi manutentivi eseguiti nel corso degli anni, l'assetto complessivo dell'edificio risente di importanti carenze strutturali, legate sia alla vetustà dell'immobile, progettato alla fine dell'Ottocento, sia alla penuria di spazi da destinare alla socialità e ad altre attività trattamentali in favore della popolazione detenuta. Giova evidenziare che, in ragione della necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui al DPR n. 230 del 2000 e di provvedere al rinnovamento completo degli impianti igienici, nonché di superare le gravi problematiche funzionali dovute alla capienza delle camere di pernottamento, è intendimento dell'amministrazione centrale avviare, già dall'anno in corso, un intervento complessivo di ristrutturazione delle sezioni detentive. Considerata l'esigenza di mantenere, nel frattempo, la funzionalità dell'istituto, seppur con capienza dimezzata, nonché di ripartire i relativi costi in più esercizi finanziari, si prevede di dividere i lavori in due lotti funzionali, uno per ciascun braccio detentivo. Pertanto, è previsto l'avvio dell'intervento di "Ristrutturazione del fabbricato detentivo, primo lotto", per un importo stimato di 2,6 milioni di euro, la cui ultimazione della progettazione definitiva - secondo il MIT - è prevista per il mese di ottobre 2024, e la conclusione della procedura di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori entro i primi mesi del 2025. Questo per il primo lotto. di Brescia Verziano, si rappresenta, in via preliminare, che, con decreto interministeriale Infrastrutture/ Giustizia del 10 ottobre 2014, è stato assentito un finanziamento di 15,2 milioni di euro per l'ampliamento dell'istituto, mediante la realizzazione di un nuovo padiglione da 340 posti. Il finanziamento, inizialmente approvato per la realizzazione dell'intera opera, nel tempo è risultato insufficiente e, nelle more dell'individuazione di fondi aggiuntivi occorrenti per il relativo completamento (38,8 milioni), è emersa la necessità di prevedere la realizzazione di un primo stralcio funzionale contemplante solo una parte dell'intervento ipotizzato in fase di fattibilità. L'amministrazione centrale, valutate le possibili ripercussioni sulla capacità ricettiva e sull'operatività dell'istituto penitenziario, connesse alla prospettata ipotesi di intervento, ha comunicato l'opportunità di dare priorità all'esecuzione del lotto funzionale concernente la realizzazione del nuovo padiglione detentivo, delle nuove centrali tecnologiche e dell'impianto di smaltimento delle acque reflue. L'ipotesi progettuale sviluppata per l'ampliamento dell'istituto di Verziano consentirà, inoltre, di mantenere adeguati spazi per l'espletamento delle fondamentali attività trattamentali in favore della popolazione detenuta. Per quanto attiene, invece, ai fondi occorrenti alla realizzazione dell'intero intervento, il MIT, in sede di riprogrammazione delle risorse finanziarie in materia di edilizia penitenziaria 2023-2030 - sottoposta all'esame del Comipa. il 6 novembre 2023 - ha previsto l'intera copertura finanziaria con previsione presuntiva di spesa complessiva dell'intervento stimata in 40,5 milioni di euro circa. Infine, quanto all'eventuale consequenziale ipotesi di dismissione, più o meno progressiva, dell'istituto di Brescia Canton Mombello, ogni analisi e determinazione in merito potrà essere eseguita solo ad ultimazione dell'intervento di ampliamento previsto previsto presso la casa di reclusione di Brescia Verziano, allorquando potranno essere più adeguatamente e correttamente valutate, in un pertinente e attuale quadro di contesto, le possibilità che la struttura sarà ancora in grado di offrire, unitamente alle contingenti esigenze detentive del relativo circondario. Nel frattempo, da informazioni acquisite dal Provveditorato regionale, è stata assegnata una somma complessiva di 291.000 euro per la corrente annualità all'istituto Canton Mombello, per la manutenzione generale della struttura. In relazione alle carenze del personale del corpo di polizia penitenziaria rispetto agli organici della casa circondariale di Brescia Canton Mombello e della casa di reclusione di Brescia Verziano, secondo i dati forniti dal DAP, alla data del 30 settembre 2024 si evince una carenza di personale impiegato comunque comune a quella risentita in tutti gli istituti penitenziari del Paese. A Canton Mombello, la forza presente, pari, allo stato, a 184 unità su un organico di 227, inferiore di 43 unità rispetto a quello previsto. Le carenze sono di 2 unità nel ruolo dei funzionari, 13 unità per il ruolo di ispettori, di 21 per i sovrintendenti, di 4 unità per il ruolo di agenti assistenti. Risulta, invece, a pieno organico il ruolo dei funzionari pedagogici. Nella casa di Brescia Verziano, la forza presente è pari, allo stato, a complessive settantasette unità su un organico di 95 unità di personale, inferiore, dunque, di 18 unità rispetto a quella prevista. Nello specifico, risultano scoperti 2 unità per funzionari, 3 ispettori, 7 sovrintendenti, mentre gli agenti assistenti sono in esubero di 2 unità. Segnalo, nello specifico, che, per quanto riguarda l'organico del ruolo dei funzionari, al fine di arginare la scopertura nel ruolo di titolare del comando di reparto, l'amministrazione centrale ha coperto la vacanza degli istituti di Brescia a partire dal 9 ottobre 2024. Come ribadito in altre occasioni in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto DAP, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace *turn over* del personale, risultando indubbie le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati. In quest'ottica, con riferimento alla carenza del ruolo di sovrintendenti, il 16 febbraio 2024 è stato bandito un ulteriore concorso interno per complessive 293 unità a copertura delle vacanze al 31 dicembre 2022. All'esito della citata procedura concorsuale, l'Amministrazione terrà conto della carenza nel ruolo sofferta dagli istituti penitenziari di Brescia con l'assegnazione di un idoneo numero di unità. Per il ruolo degli ispettori, nel mese di novembre si è concluso il VII corso ispettori e si segnala che alla casa circondariale di Brescia Canton Mombello, in particolare, sono state assegnate 4 unità maschili. Per quanto riguarda il ruolo degli agenti-assistenti, l'organico della casa circondariale di Brescia Canton Mombello è stato incrementato, di recente, di 6 unità maschili e di 3 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria. Affrontando, infine, il problema delle presenze detentive, alla data del 25 giugno 2024, presso la casa circondariale di Brescia Canton Mombello sono presenti 377 detenuti, rispetto a una capienza di 182 posti, con una percentuale di affollamento pari al 207,14 per cento. L'emergenza è chiara e prioritaria, tanto che, con iniziative di contrasto al sovraffollamento carcerario, la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha proseguito l'opera di riequilibrio della popolazione detentiva su territorio nazionale mediante l'emissione, per la sola Regione Lombardia, di ulteriori otto provvedimenti deflattivi per un totale di 141 detenuti, operando un costante monitoraggio delle presenze. Si confida chiaramente in un significativo abbattimento della percentuale riportata anche alla luce degli importanti interventi di edificazione e ristrutturazione che ho qui illustrato. Non si dimentichi, infine, che le direttrici su cui il Governo sta costantemente lavorando sono molteplici e complesse. La normativa di recente approvazione, infatti, oltre all'ampliamento della capacità ricettiva degli istituti penitenziari, è orientata, in generale, a umanizzare l'esecuzione della pena, favorendo il ricorso a misure alternative alla detenzione, prevedendo la limitazione della carcerazione preventiva, il trasferimento di minori e tossicodipendenti nelle apposite comunità, l'ampliamento e il rafforzamento delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale.

e ha avuto un impatto nullo sulla situazione attuale: erano 61.300 i detenuti a fine luglio e adesso ne sono 61.700; quindi, dal punto di vista della capacità deflattiva della popolazione carceraria, l'impatto di quel decreto è stato nullo.

e pensare di risolvere la questione semplicemente attraverso la costruzione di nuovi padiglioni per i quali ci vorranno anni vuol dire non affrontare l'emergenza. Siamo altresì preoccupati per il fatto che, a dispetto delle parole che vengono spese ogni volta che si parla della questione, le politiche della giustizia di questo Governo vanno in direzione diametralmente opposta.

farà il paio con quanto è accaduto con il decreto Caivano: proprio nei giorni scorsi l'associazione Antigone ha lanciato il grido d'allarme sugli istituti penitenziari minorili italiani, che sono sempre stati un fiore all'occhiello del nostro sistema giudiziario; dopo quel decreto c'è stato infatti un aumento esponenziale della popolazione carceraria negli istituti minorili, con effetti disastrosi dal punto di vista del trattamento educativo e rieducativo dei minori ivi detenuti, e le numerose rivolte che stanno scoppiando in quegli istituti penitenziari segnalano quanto la situazione sia drammatica. Devo dire che ci saremmo aspettati, dopo l'improvvisa morte del compianto onorevole D'Ettore come garante dei detenuti, dei detenuti, un maggior coinvolgimento anche del Parlamento e delle opposizioni nei criteri di valutazione delle scelte del nuovo garante. Proprio in questo momento un garante efficace e presente è molto importante per monitorare le condizioni dei nostri penitenziari. E la scelta, ricaduta invece su una

al controllato, non garantisce rispetto ai requisiti di indipendenza e di autonomia che un garante dei detenuti dovrebbe avere. Ma vengo al tema del carcere di Brescia Canton Mombello, che è paradigmatico della condizione generale. Lei ha citato i numeri: 380 detenuti su una capienza ordinaria di 180 posti.

e siamo ancora alle prese con la necessità di avviare i lavori. Prendiamo atto del fatto che c'è la volontà di proseguire, però invitiamo davvero l'Amministrazione a fare il possibile, perché la condizione attuale è inaccettabile. è inaccettabile il fatto che si pensi di spendere 40 milioni di euro per un nuovo padiglione senza avere ancora chiara la necessità di chiudere l'attuale carcere, che non può essere ristrutturato, perché assolutamente inadeguato alle funzioni rieducative e trattamentali di un penitenziario moderno. Prendo quindi atto della volontà del Governo di continuare a perseguire quest'opera strategica, ma invito ad accelerare i tempi, perché la situazione è veramente inaccettabile per una città di grande civiltà come Brescia.

Al riguardo, in via preliminare ricordo che il carattere di ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, è disciplinato dal decreto-legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma e trova un utile riferimento nelle disposizioni di cui al testo unico delle imposte sui redditi concernenti la determinazione del reddito degli agricoltori. Con riguardo all'ISEE, è opportuno premettere che, ai sensi del DPCM n. 159 del 2013, esso è determinato mediante una scala di equivalenza in funzione della composizione del nucleo familiare e ha riguardo al reddito, nonché al patrimonio di tutti i suoi componenti. Evidenzio inoltre che le componenti di natura reddituale e patrimoniale nell'ISEE costituiscono elementi dell'indicatore distintamente considerati. Tanto chiarito e con specifico riferimento alla componente riferita al patrimonio immobiliare, giova richiamare l'articolo 5, comma 2, del citato DPCM, secondo cui il il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercitanti l'attività di impresa, quale definito ai fini dell'IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione del pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, Grazie per mutui contratti nell'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Questa è la parte del riferimento normativo. Alla luce del quadro normativo sopra illustrato, è stato poi esaminato, nell'ambito del tavolo tecnico composto dalla Consulta nazionale dei centri assistenza fiscale (CAF), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Agenzia delle entrate e anche dall'INPS, il tema dell'inserimento dei fabbricati rurali nella dichiarazione sostitutiva unica. Rispondendo quindi allo specifico quesito posto dall'interrogante, evidenzio che, in linea generale, i fabbricati rurali devono essere autodichiarati nel quadro FC3 della DSU, relativo al patrimonio immobiliare, con le seguenti peculiarità ed eccezioni in funzione della fattispecie concreta; i fabbricati rurali che non hanno un valore ai fini IMU sono inclusi nel valore del terreno, oppure gli immobili strumentali all'attività non vanno dichiarati nel quadro FC3, ma contribuiscono al patrimonio netto dell'impresa nel quadro CF2, CF2, sezione II, della dichiarazione concernente la valorizzazione del patrimonio mobiliare. Rappresento che il suddetto chiarimento è stato inserito quale informazione prontamente e generalmente fruibile in una FAQ pubblicata il 13 settembre ultimo scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel portale unico ISEE dell'INPS. Siamo ben consapevoli che l'ISEE condiziona l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e, proprio per questo motivo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato impulso all'attività di revisione del regolamento ISEE, risalente al 2013, che sino ad oggi non era mai stato aggiornato, avviando il necessario confronto con le amministrazioni interessate. A seguito dell'introduzione della previsione relativa all'esclusione dei titoli di Stato nella determinazione dell'ISEE, nella legge di bilancio 2024 si è predisposto uno schema di DPCM, in corso di definizione, che, oltre a recepire le modifiche normative apportate nel tempo dalla disciplina ISEE, dà attuazione alla citata disposizione di cui all'articolo 1,

Grazie al dialogo e al confronto con il Parlamento, il Governo continuerà a lavorare in sinergia per individuare le criticità, tradurle in aree di intervento e riflettere sulle soluzioni perseguibili con la consueta dedizione, considerando ovviamente prioritaria tale azione di governo in quanto risponde ad esigenze sociali e quindi a risposte fondamentali

Grazie Bellucci per la ricostruzione e prendo atto della risposta fornita, che ovviamente va studiata in dettaglio anche per quel che riguarda la FAQ da lei da lei citata. Ritengo comunque che sia ora di fare chiarezza sulla questione. Si tratta infatti di una questione importante. Sappiamo tutti che l'ISEE è l'indicatore che determina le condizioni economiche del nucleo familiare al fine dell'accesso a determinati servizi e alle agevolazioni socioassistenziali e, quindi, fa una enorme differenza ricomprendere o meno nella determinazione dell'ISEE i fabbricati rurali in uso all'imprenditore agricolo per svolgere la propria attività di agricoltore. Ringrazio molto anche per aver fornito la risposta Grazie

Presidente, ringrazio l'interrogante e risponderò a questa interrogazione per quanto di ragione e per quello che è di stretta competenza del Ministero della giustizia. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, segnalo che, in seguito alla cessazione degli effetti dei contratti di digitalizzazione dei fascicoli negli uffici giudiziari italiani - ripeto: cessazione degli effetti - la competente articolazione del Ministero, per il tramite dei preposti uffici, ha indetto una nuova gara. Il servizio è stato suddiviso in cinque lotti e precisamente: CISIA Milano, CISIA Bologna, CISIA Roma, CISIA Napoli e CISIA Palermo. La suddivisione è stata effettuata seguendo l'articolazione degli uffici dirigenziali non generali di coordinamento interdistrettuale. Per l'espletamento della gara, trattandosi di contratti con valore superiore alla soglia europea, si è ritenuto di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con una remunerazione del personale ancorata al criterio delle pagine scansionate. Elenco di seguito lo stato attuale delle gare relative ai cinque lotti e ripeto per quanto di stretta competenza del Ministero che qui rappresento. CISIA di Bologna: la gara è stata aggiudicata al fornitore Datamanagement Italia SpA, il contratto è stato firmato, i controlli riservati agli organi contabili hanno avuto esito positivo ed è stata avviata l'esecuzione. CISIA di Milano: la gara è stata aggiudicata al fornitore di Datamanagement Italia SpA, il contratto è stato firmato, i controlli riservati agli organi contabili hanno avuto esito positivo ed è stata avviata l'esecuzione. CISIA di Napoli: la gara è stata aggiudicata al fornitore Datamanagement Italia SpA, il contratto non è stato ancora sottoscritto, pende infatti un ricorso innanzi al TAR della Campania ed è stata fissata l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare per il prossimo 9 ottobre 2024. CISIA di Palermo: la gara è stata aggiudicata al fornitore Datamanagement Italia SpA, il contratto è stato firmato, i controlli riservati agli organi contabili hanno avuto esito positivo ed è stata avviata l'esecuzione. CISIA di Roma: la gara è stata aggiudicata al fornitore ISPAR Srl, il contratto non è stato ancora sottoscritto, pende innanzi al TAR del Lazio un'impugnativa dell'esito della gara pubblica. Tengo a sottolineare che su tutti i soggetti aggiudicatari sono stati eseguiti i controlli prescritti dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice degli appalti pubblici). Lo scorso 5 agosto 2024 la competente direzione del Ministero della giustizia ha disposto, a prescindere dalle impugnazioni degli esiti delle gare pubbliche, l'esecuzione anticipata di tutte le attività contrattuali, ai sensi dell'articolo 17 del codice degli appalti, per rispettare le scadenze imposte dalla *milestone* M1C1-153 del PNRR in tema di digitalizzazione degli atti processuali e per evitare una sospensione prolungata del servizio di digitalizzazione degli stessi negli uffici giudiziari italiani. Grazie VERINI *(PD-IDP)*. Vice Ministro, la ringraziamo per la risposta, che tuttavia ci pare un po' burocratica. Noi abbiamo posto con questa interrogazione, sia qui, sia precedentemente e analogamente alla Camera, alcuni problemi che riguardano un servizio importante, quello della digitalizzazione del processo penale telematico, una delle strade più importanti

ancora molta è la fatica da sopportare. Quando si parla di queste cose, si deve tenere a cuore la funzionalità del servizio, perché noi siamo per una giustizia che funzioni e per una ragionevole durata dei processi, anche se riconosco che l'applicazione rigida del processo telematico al penale va contemperata con le esigenze, a volte, di presenza fisica dell'imputato o degli imputati, per esercitare nel pieno il diritto di difesa. A parte questo stupisce che il Ministero, nel momento in cui decide di fare un bando, poi non segua da vicino l'*iter* del bando stesso. Di fatto in questa procedura è stato violato almeno un paio di volte il contenuto del nuovo codice degli appalti, che pure ha già allentato di molto le tutele dei lavoratori, le tutele delle imprese e la sicurezza nel lavoro.

l'obiettivo di garantire comunque il rispetto dei contratti di lavoro e la sicurezza del posto di lavoro. In questo caso tutto ciò non c'è stato; ci sono state professionalità consolidate, famiglie e diciotto dipendenti di un servizio di fatto sono stati mortificati. Nel nuovo codice si prevede che in certi casi ci sia una sorta di contrattazione-dialogo con i sindacati per servizi importanti che riguardano, per esempio, la procura di Roma, quelle del Lazio e di altre Regioni limitrofe; si tratta di servizi delicati. Non c'è stato alcun coinvolgimento, ed ecco perché non ci dichiariamo soddisfatti della sua risposta.

abbiamo lavorato molto insieme nella scorsa legislatura. Ci sono stati dei Governi, in particolare l'ultimo, quello guidato da Mario Draghi con il ministro Cartabia, che hanno proceduto a delle riforme di sistema, certamente perfettibili perché erano comunque fatte anche da una maggioranza molto ampia, ma che secondo noi avrebbero dovuto essere applicate. Voi avete scelto una strada diversa, quella di disarticolarle, di mettere in discussione quello che si era fatto senza legiferare contro qualcuno o a favore di qualcuno, ma con riforme che avevano un obiettivo, ossia l'efficienza del processo penale, l'efficienza del processo civile, una riforma dell'ordinamento. Voi avete capovolto: avete rimesso l'elmetto, avete ridichiarato guerra alla magistratura e avete introdotto e state introducendo elementi divisivi. Il punto della strada che avete scelto però qual è, oltre che - secondo noi - essere molto sbagliata? Non vi occupate del funzionamento reale e quotidiano degli uffici giudiziari, e questo episodio ne è un altro esempio.

Come è noto, la procedura di pagamento degli stipendi del personale supplente breve e saltuario risulta piuttosto complessa a causa dei vincoli amministrativi e normativi che richiedono adempimenti e controlli da parte di diverse amministrazioni. L'attuale processo di pagamento prevede che l'inserimento dei contratti, le eventuali variazioni dello stato giuridico e l'autorizzazione dei ratei siano compiti delle istituzioni scolastiche, mentre l'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole è di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. L'elaborazione del cedolino unico e la liquidazione dei compensi spettano invece al Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, il corretto completamento della procedura dipende dal rispetto degli adempimenti previsti nelle fasi sopra descritte e dalle tempistiche indicate nel DPCM del 31 agosto 2016, relativo al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Alla luce di ciò, durante il 2023, in seguito all'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021, la liquidazione degli arretrati dovuti ai contratti di supplenza breve e saltuaria ha comportato una riduzione delle risorse finanziarie allocate sui capitoli pertinenti. Per far fronte a questa situazione, il Ministero dell'istruzione e del merito si è tempestivamente attivato presso il MEF per reperire le risorse finanziarie necessarie e apportare le opportune variazioni di bilancio al fine di ripristinare le disponibilità sui suddetti capitoli. È importante sottolineare che - come già avvenuto negli anni finanziari precedenti anche per il 2023 il Ministero ha identificato ulteriori economie sui capitoli relativi agli incarichi aggiuntivi (Covid), pari a 55,6 milioni di euro. Grazie a una specifica disposizione legislativa, tali risorse sono state destinate all'incremento dei capitoli relativi alle supplenze brevi e saltuarie (articolo 10, comma 2, del Inoltre, con l'emissione straordinaria di gennaio 2024, richiesta dal Ministero a NoiPA, sono stati effettuati i pagamenti dei ratei non ancora coperti, oltre agli emolumenti di dicembre non ancora retribuiti, per un totale di circa 300 milioni di euro. A partire dall'8 gennaio 2024, sono state anche predisposte due assegnazioni mensili per coprire il fabbisogno relativo ai contratti di supplenza breve e saltuaria. Queste iniziative hanno permesso di saldare sia i ratei stipendiali arretrati, che quelli relativi ai nuovi contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche. Infine, per fronteggiare il fabbisogno finanziario

richieste dall'amministrazione nella legge di assestamento di bilancio, pari a poco più di 152 milioni di euro lordi. Ciò consentirà di gestire con maggiore tranquillità le assegnazioni dei prossimi mesi. Vorrei inoltre sottolineare che, su impulso del ministro Valditara, è stato intensificato il coordinamento con il MEF e NoiPA, con l'obiettivo di riformare in maniera organica e strutturale la procedura di pagamento. Meloni, le misure finora attuate hanno permesso non solo il pagamento dei ratei contrattuali dei periodi pregressi, ma anche il riallineamento della maggior parte delle retribuzioni, mitigando significativamente le criticità segnalate.

trovo questa risposta piuttosto deludente. Il ministro Valditara aveva annunciato all'inizio del 2023, presentando le sue linee programmatiche, che le riforme delle procedure, di cui lei ci ha parlato anche ora, sarebbero state attuate. Ha parlato di 20 misure, tra cui rientrava anche la riduzione dei tempi dei pagamenti del personale supplente.

funzioni senza che le persone possano operarvi in termini adeguati a corrispondere a un'esigenza che è semplicemente consentire a persone che

di rendere le modalità di pagamento per il personale per supplenze brevi e saltuarie simili a quelle per il personale supplente in maternità. A quanto ci consta, non è stato avviato alcun tipo di confronto e non è stata presa in considerazione la richiesta dei sindacati. Tutto questo avviene in un contesto nel quale, negli ultimi sette anni, i docenti precari sono aumentati di oltre il 70 per cento: lo scorso anno sono stati oltre 230.000 e quest'anno dovrebbero essere 250.000. In tale contesto non si comprende e non sappiamo una cosa. Chiediamo che ne è degli idonei del concorso straordinario del 2020, che sono ancora lì, senza un vostro intervento che ne faciliti l'ingresso tra il personale strutturato. Abbiamo ancora problemi

cento (mentre negli altri Paesi gli stipendi sono aumentati del 4 per cento). In questo contesto voi continuate a tagliare sull'istruzione: tagli di 500 milioni nella vostra prima legge di bilancio, tagli di 100 milioni nella scorsa legge di bilancio per il 2024 e nessun nuovo investimento. Di tanto in tanto dite che intervenite sull'edilizia, sugli asili, sui rinnovi dei contratti. Sarebbe più onesto dire che queste sono risorse PNRR che derivano da un'iniziativa politica, da atti politici e parlamentari che provengono dal centrosinistra. Va bene che utilizziate queste risorse, ma il fatto che non investiate nessuna nuova risorsa sull'istruzione è una responsabilità pesantissima pesantissima che questo Governo ha sulle spalle e credo che la sua risposta - che ci dice che effettivamente le persone che lavorano prima o poi devono essere pagate - sia davvero deludente.

Presidente, è in corso lo svolgimento delle interrogazioni e quindi sono presenti il Governo e soltanto i senatori interroganti.

Signor Presidente, ringrazio il senatore Parrini per il quesito posto, concernente le vicende relative alla collocazione del dipinto della Visitazione del Pontormo, che a breve sarà nuovamente esposto al pubblico nella Villa medicea di Poggio a Caiano, in provincia di Prato. In realtà l'inaugurazione era in programma proprio oggi, ma è stata posticipata per via dell'allerta meteorologica L'opera della Visitazione era ospitata nella chiesa di San Michele Arcangelo e San Francesco in Carmignano in quanto di proprietà della relativa parrocchia. Tale sito religioso, nel 2023, è stato chiuso al pubblico a causa di infiltrazioni d'acqua delle coperture che ne hanno determinato l'inagibilità, come constatato nel sopralluogo effettuato dalla soprintendenza territorialmente competente agli inizi dello scorso novembre. I tecnici incaricati dalla parrocchia riferiscono altresì che al precario stato della chiesa si aggiungono rischi strutturali che interessano le capriate. Da qui la necessità di lavori nell'aula della chiesa, oltre a quelli da effettuare nelle altre parti del convento che hanno subito crolli estesi. La Visitazione si presenta oggi in buono stato e, tra l'altro, è stata restaurata di recente. Inoltre, trattandosi di un'opera dipinta su tavola, richiede condizioni sicure e controllate di umidità e temperatura. Pertanto, la sovrintendenza ha dato disposizioni alla parrocchia di mettere in sicurezza le opere presenti nella chiesa, tra cui appunto la Visitazione, e di attivarsi per trovare una diversa collocazione temporanea. La diocesi di Pistoia ha accolto la proposta avanzata dal Comune di Poggio a Caiano e dalla direzione regionale musei della Toscana, di esporre la Visitazione del Pontormo presso la Villa medicea di Poggio a Caiano e gli altri sei dipinti presso la Sala della giostra del Palazzo comunale. Detta scelta è stata adottata, tra l'altro, tenendo conto della vicinanza territoriale e tematica dell'opera, data la presenza di alcuni affreschi del Pontormo nel medesimo territorio, così da creare un diretto dialogo fra le opere. Il 3 maggio 2024, il Comune di Poggio a Caiano, il Comune di Carmignano, la direzione regionale musei della Toscana e la parrocchia di San Michele Arcangelo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il quale hanno stabilito la presa in carico e il trasporto assicurato delle opere; la collocazione nelle sedi temporanee e relativo allestimento; la custodia, la promozione e valorizzazione, la ricollocazione nella sede originaria al termine dei lavori nella chiesa di San Michele Arcangelo e San Francesco in Carmignano. Sulla base di detto protocollo, la direzione regionale musei della Toscana si è assunta l'onere della custodia e conservazione della Visitazione all'interno del museo statale Villa medicea sulla base di un comodato con la parrocchia e l'impegno ad attivare la garanzia di Stato a copertura della giacenza dell'opera nel museo. Il protocollo della durata di cinque anni rinnovabili ha anche la finalità di ricollocare le opere nella sede originaria al termine dei lavori nella chiesa. Così, a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa, la Visitazione è stata collocata nella Villa medicea e le altre opere nella Sala della giostra. Si fa presente che la direzione generale musei ha inoltre stanziato un finanziamento di 35.000 euro a favore della direzione regionale musei nazionali della Toscana per poter procedere in tempi brevi a tutte le operazioni legate all'allestimento della Visitazione, nella sala appunto della villa di Poggio a Caiano, e all'adeguamento delle condizioni microclimatiche della stessa. Il Ministero della cultura si impegnerà fattivamente al fine di poter contribuire al ripristino della chiesa di San Michele Arcangelo e San Francesco in Carmignano, affinché l'opera del Pontormo possa ritornare nella sua sede propria.

il protocollo cui ha fatto riferimento nella parte finale dell'intervento esplicita l'obiettivo finale, quello di far tornare la Visitazione di Pontormo, una delle opere magnifiche del Carucci, dove è stata per secoli e dove dovrà rimanere per i secoli a venire, ossia a Carmignano. Presso molti critici d'arte quest'opera è conosciuta come la Visitazione di Carmignano e non è immaginabile che possa stare altrove. La delusione deriva dal fatto che, accanto all'indicazione di questo obiettivo finale (meno male che c'è), non c'è però la risposta al quesito principale della mia interrogazione. Io chiedevo che cosa il Ministero stia facendo per mettere a disposizione i 600.000 euro che servono per i lavori nella chiesa di Carmignano, affinché questa possa tornare in possesso di un'opera che è legittimo e giusto che stia lì e che non può stare altrove, altrimenti la comunità di Carmignano si sentirebbe vittima quasi di uno scippo civile. Purtroppo su questo non mi pare che il Sottosegretario sia stato in grado di fornire alcuna certezza e credo sia un punto dolente. Ho il massimo apprezzamento, anche per aver fatto il sindaco in un Comune vicino, per i Comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano, per la qualità e la bellezza della Villa medicea di Poggio a Caiano. Resta il fatto che c'è una ferita da chiudere. C'è una comunità, quella di Carmignano, che per secoli ha avuto un'opera importantissima, che adesso non può più averla sul proprio territorio e che, per tornare ad averla, chiede allo Stato di impegnare non 60 o 6 milioni di euro, ma alcune centinaia di migliaia di euro e questo va fatto al più presto. Mi auguro che le certezze che oggi non sono state date possano essere date velocemente possano essere date velocemente ai cittadini di Carmignano e a tutti i cittadini toscani, ammiratori del Pontormo, estimatori dell'arte cinquecentesca e, in generale, amanti della cultura, che si aspettano che questa ferita possa essere chiusa.

alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

è il Presidente di turno del G7 in un 2024 segnato da rilevanti fatti di politica internazionale cui facciamo riferimento nella nostra nota. L'Ucraina, il Medio Oriente - lo vediamo in queste ore - l'Africa, di cui noi parliamo poco, ma di cui Russia e Cina parlano - anzi, fanno - molto. La nostra impressione è che l'Italia, nella Presidenza del G7 esteri, non abbia brillato: che lei, signor Ministro, non abbia brillato. Non ricordiamo una idea, una proposta che, sotto la sua Presidenza, in questo 2024 così complesso, abbiamo non dico portato a casa, ma neanche messo sul tavolo.

che sulla politica estera rileva il giusto, ma sulla politica interna, come Vice Presidente, lei ha messo in campo, cioè lo *ius scholae* - e noi siamo d'accordo con lei - le chiedo se dobbiamo credere al Tajani di agosto, che è per il sì allo *ius scholae*, o alla versione aggiornata del Tajani di settembre, che è per il sì a Salvini e Meloni e per il no allo *ius scholae*, così almeno capiamo di cosa si occupava in questi mesi il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri.

agli interroganti sulla questione della politica internazionale, e non sulla politica interna. Si è chiesto come siamo collocati. A livello internazionale la posizione del Governo è chiara e inequivocabile: europeismo e atlantismo sono le stelle polari della nostra politica estera. L'appartenenza all'Unione europea, all'Alleanza atlantica e il rapporto di forte amicizia con gli Stati Uniti sono alla base di tutte le nostre scelte strategiche e guidano la nostra azione di fronte alle principali sfide che stiamo affrontando in questa fase storica, particolarmente complessa. Il nostro Governo può rivendicare con orgoglio di essere sempre stato in prima linea al fianco dell'Ucraina: il sostegno a Kiev, alla sua libertà, indipendenza e sovranità è pieno e incondizionato. Proprio in quest'ottica ho voluto co-presiedere a New York, con il segretario di Stato Blinken e il nuovo ministro degli esteri ucraino Sybiha, una sessione speciale del G7 a sostegno del settore energetico ucraino. Abbiamo concordato una serie di ulteriori misure a sostegno della popolazione civile per far fronte ai bisogni più immediati, anche in vista dell'arrivo dell'inverno. Ho valorizzato in tal senso i fondi stanziati dal Governo, il contributo delle aziende italiane e l'accordo che abbiamo concluso con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - li ho firmati con il Ministro precedente - prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro per ripristinare la capacità della principale società idroelettrica ucraina. Questo è stato fatto dalla Presidenza italiana del G7. Il disegno di legge di ratifica è stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 30 agosto ed è ora all'esame del Parlamento per quella che auspico sarà una rapida approvazione, e mi auguro anche con il sostegno dell'interrogante. In ambito G7 tutti hanno apprezzato l'impegno del Governo italiano per la ricostruzione, come testimoniato anche dall'importante conferenza internazionale che ospiteremo nel 2025. Vorrei annunciare sin d'ora che stiamo lavorando per coinvolgere il Parlamento in una specifica sessione dei lavori di quella conferenza. Sosteniamo Kiev senza se e senza ma anche dal punto di vista politico e militare, come ho ribadito anche nel mio recente intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Abbiamo approvato nove pacchetti di sostegno militare per difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina, in coordinamento con gli alleati della NATO e dell'Unione europea. Mi fa piacere informare il senatore interrogante che, durante la riunione del Consiglio europeo affari esteri, l'Alto rappresentante ha proposto di abolire qualsiasi limitazione all'uso delle armi che diamo all'Ucraina. Il Consiglio affari esteri non ha approvato la proposta dell'alto rappresentante Borrell. Quindi, l'Italia non è assolutamente isolata e non risponde a verità ciò che l'interrogante abbiamo approvato nove pacchetti a sostegno militare, quindi è un sostegno a 360 gradi, apprezzato da Kiev e riconosciuto da tutti i nostri *partner.* Anche sul Medio Oriente la nostra posizione è molto chiara: lavoriamo in stretto coordinamento con i nostri principali alleati e con i partner regionali. Gli obiettivi che ho ribadito anche ieri nella riunione del Quintetto (Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) sono i seguenti: cessate il fuoco a Gaza e in Libano; nuovi aiuti umanitari alla popolazione civile; ripresa di percorsi negoziali per la stabilizzazione del confine israelo-palestinese; di uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. Il nostro Governo resta impegnato come Presidenza del G7 in seno al quintetto, alle Nazioni Unite e all'Unione europea per favorire il dialogo e contribuire alla pace. E continueremo a lavorare in questa direzione con la forza di una politica estera che ha ben chiari i propri valori, la propria identità e l'interesse del Paese che questo Governo ha l'onore di rappresentare. nuova finestra") *(IV-C-RE)*. Signor Ministro, non ci ha convinto, ma non è una novità e non è neanche una sorpresa, al netto di un particolare su cui lo smentisco. Ella ha detto che io mi sarei confuso sulla solitudine, ma ho fatto riferimento al fatto che l'Italia è l'unico Paese del G7 che ha

dell'Iran su Israele, lei postava il seguente *tweet:* «Benvenuta alla consigliera regionale Linda Elezi, eletta nel collegio della Provincia di Ancona.

per andare a visitare l'Africa subsahariana probabilmente aspetterà che si apra una sezione di Forza Italia in Congo o in Namibia, e così finalmente ci va. È l'unico che non ci è mai andato, ci manda la Meloni e meno male che ci va lei. Quanto alla battutina iniziale - e termino restando nei due minuti

il Tajani di settembre ha detto che non lo avrebbero votato perché Meloni e Salvini non volevano. Abbiamo inaugurato la versione del Tajani di ottobre. Non è il Tajani del sì di agosto, non è il Tajani del no di settembre: è il Tajani del boh. Buon ottobre anche a lei, signor Ministro.

una risposta che stia sul tema; non ci faremo certo dettare l'agenda da provocazioni che sanno più di campagna elettorale che non di serietà rispetto al momento che stiamo vivendo. *(Applausi)*. Nessuno di noi, signor Ministro, può dimenticare il brutale attacco di un anno fa, il 7 ottobre 2023. Quell'attacco ha riacceso le tensioni, alimentato nuovi focolai di conflitto nella regione e negli ultimi giorni, purtroppo, il conflitto si è allargato - questa è la sostanza delle cose anche sul fronte libanese, dove lo Stato di Israele ha intensificato le operazioni militari in risposta alle minacce e agli attacchi provenienti dal movimento sciita di Hezbollah. L'attacco missilistico lanciato dall'Iran contro Israele ha reso ancora più urgente intensificare gli sforzi per fermare la spirale di violenza e raggiungere un cessate il fuoco. L'*escalation* del conflitto tra Israele e Hezbollah ha già avuto un impatto molto pesante sulla popolazione civile e nelle aree più colpite decine di migliaia di persone hanno lasciato le loro abitazioni per dirigersi verso altre aree ritenute più sicure, nel più ampio movimento di popolazione dal conflitto del 2006. Il Governo italiano, anche in qualità di Presidenza del G7, si sta adoperando con i *partner* internazionali e regionali per sostenere gli sforzi di mediazione in corso e noi siamo grati a lei e al presidente Meloni, perché sappiamo quanto sia importante la presenza dell'Italia a quei tavoli e quanto sia apprezzata e invocata. È bene quindi che si lavori con il nostro comune sentire e che l'Italia ci sia. Le chiediamo, signor Ministro, quali ulteriori iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere anche in ambito G7 e Quint, a cui lei faceva riferimento, dal quale ci aspettiamo anche davvero posizioni forti, al fine di tentare di contenere la nuova *escalation*

mi permetta di esprimere il mio sconcerto per l'atteggiamento del precedente interrogante che ha così grande interesse per la politica estera che, appena ha parlato, se ne è andato comunque che il giudizio sulla sua politica e su quella che faccio io l'abbiano dato gli elettori in occasione delle elezioni europee. Rispondo subito all'onorevole Paroli. L'*escalation* del conflitto tra Israele e Hezbollah… Lasciate intervenire il Ministro. Senatore Lorefice, ci sono io che sto presiedendo, se non le dispiace. Prego, Ministro, vada pure avanti. L'*escalation* del conflitto tra Israele e Hezbollah ha già avuto un impatto molto pesante sulla popolazione civile. È necessaria una risposta umanitaria rapida e incisiva, soprattutto a fronte della situazione degli sfollati, la più grave dal conflitto del 2006. A tal riguardo, vorrei fare subito un annuncio in anteprima qui nell'Aula del Senato. Ho deciso di aprire il G7 Sviluppo di Pescara del 22 ottobre con una Conferenza internazionale umanitaria sul Medio Oriente, per far fronte in particolare alla difficile situazione in Libano e a Gaza. *(Applausi)*. Saranno presenti le agenzie delle Nazioni Unite, la società civile e le associazioni di categoria. Ne parlerò tra poco anche con l'alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi. Valorizzeremo che sul fronte umanitario siamo stati i primi a muoverci. Lo abbiamo fatto varando un nuovo importante pacchetto di aiuti (17 milioni) dedicati alla crisi libanese, che si aggiungono ai 50 milioni già stanziati. L'apertura del fronte libanese e il nuovo intervento diretto dell'Iran aumentano significativamente il rischio di un conflitto regionale su vasta scala. Il Governo italiano si sta adoperando a tutti i livelli per scongiurare questo scenario. Ieri il Presidente del Consiglio ha presieduto una riunione del G7 a seguito dell'aggravarsi della crisi. I *leader* hanno ribadito la ferma condanna all'attacco iraniano e confermato l'impegno comune a favorire la riduzione delle tensioni a livello regionale. Ne ho parlato ieri anche con i Ministri degli esteri dei Paesi del quintetto (Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania). Ho illustrato i cinque punti già evidenziati nella riunione del Consiglio affari esteri straordinario di lunedì scorso: primo, insistere per un cessate il fuoco; secondo, rafforzare il mandato di UNIFIL e proteggere i militari italiani; terzo, raggiungere un accordo politico in Libano per l'elezione del nuovo Presidente; quarto, coordinare a livello europeo il rientro dei cittadini; quinto, rafforzare l'aiuto umanitario a favore della popolazione libanese. Ciò che è successo a Gaza non può ripetersi anche in Libano. È essenziale assicurare la protezione dei civili, per evitare che le ostilità possano avere lo stesso altissimo costo in termini di vite umane di un anno di guerra nella Striscia. La *de-escalation* non è solo una necessità umanitaria, ma è anche una condizione essenziale per riportare l'intero quadrante su un cammino di dialogo e stabilità. È un percorso complesso, ma è un risultato che possiamo ottenere con l'impegno e la responsabilità di tutti gli attori coinvolti. Lavoriamo affinché anche l'iniziativa umanitaria del G7 di Pescara rappresenti un tassello qualificante di questo processo.

un'accoglienza e una tutela all'interno dei tavoli che devono continuare a lavorare per la pace. Ringrazio lei e il Governo per l'importante lavoro che state svolgendo per la pace e per il dialogo. C'è ancora la possibilità di scongiurare una guerra che coinvolga l'intero Medio Oriente. Bene fa lei e bene fa la presidente Meloni a ricordarlo continuamente, perché guai se si perdesse la speranza che questo possa ancora accadere. Condividiamo l'appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali. Serve che ci sia davvero una condivisione di questo intento e troviamo sia fondamentale tenere vivo il negoziato, sostenendo, nel ruolo che ora ha l'Italia di Presidente del G7 giustamente anche all'interno del quintetto, gli sforzi di mediazione che gli Stati Uniti stanno compiendo insieme all'Egitto e al Qatar. È indispensabile che si lavori tutti insieme e che tutti i canali di comunicazione a disposizione, compresi quelli con l'Iran e con i Paesi arabi moderati, vengano attivati, così come sta facendo. Dichiarando la nostra assoluta soddisfazione per la sua risposta, voglio anche aggiungere che siamo innanzitutto soddisfatti del suo lavoro. Grazie e speriamo che prevalgano la pace e il dialogo.

cioè avvenendo quello che tutti noi, a parole, avevamo detto che non doveva avvenire, ossia una *escalation* senza fine. Appare quindi adesso il momento di uno scatto e di un impegno maggiore. Ieri abbiamo visto il comunicato del G7, che noi riteniamo tardivo perché bisognava

quelle sul Libano, sia quelle che riguardano uno Stato palestinese, sia quelle che riguardano la sicurezza di Israele. Noi non siamo equidistanti, siamo equivicini ai due popoli. Ci pare che questo sia il momento per la diplomazia italiana di riprendere in mano un filo di maggiore incisività e di maggiore qualità, perché quello che accade nel Mediterraneo è essenzialmente un problema nostro. Signor Ministro, non siamo qui per siamo qui per aiutarla e per aiutare il Governo; ci riconosciamo se il Governo rimane nel solco della tradizione diplomatica italiana, ma vorremmo capire se veramente questo salto di qualità è alle porte o se dobbiamo ancora attendere gli appelli politici

Il Governo italiano, anche in qualità di Presidente del G7, si sta adoperando ad ogni livello per raggiungere questo obiettivo e per la tutela dei connazionali nella regione e dei nostri militari in Libano. La nostra prima preoccupazione, come illustrato ieri di fronte alle Commissioni parlamentari difesa e esteri di Camera e Senato, è la loro sicurezza. In una situazione sul terreno particolarmente complessa, ci stiamo adoperando per favorire un aumento dei collegamenti in uscita da Beirut, inclusi i voli *charter* e altre modalità su cui lavoriamo con il Ministero della difesa. Proprio in queste ore stiamo organizzando un volo *charter* speciale per trasferire in Italia circa 180 connazionali, che speriamo possano arrivare già in serata. Agli italiani in Iran, circa 700, abbiamo anche raccomandato di tornare in Italia con i voli commerciali che sono in graduale ripresa. L'unità di crisi della Farnesina e le nostre ambasciate a Beirut, a Teheran e a Tel Aviv e il consolato generale a Gerusalemme lavorano senza sosta per offrire costanti aggiornamenti di sicurezza e ogni possibile assistenza. I focolai in atto riguardano ormai un quadrante molto vasto e sono tra loro interconnessi. Epicentro della crisi è ora il Libano. La soluzione diplomatica ruota anche intorno al rafforzamento della capacità operativa di UNIFIL, che abbiamo richiesto da tempo, anche in occasione del Consiglio europeo affari esteri, e che deve essere messa nelle condizioni di svolgere appieno il suo mandato. Tuttavia, non dipende da noi, ma dipende dalle Nazioni Unite prendere questa decisione, perché il Governo italiano non è il Governo che decide i destini del Medio Oriente, del Mediterraneo e del mondo intero. Siamo un Paese importante, ma quello che non riescono a fare gli Stati Uniti, la Cina e la Russia non credo che lo possa fare l'Italia da sola. Stiamo

La soluzione diplomatica, come dicevo, ruota attorno a questo rafforzamento della capacità di UNIFIL, che deve essere messa nelle condizioni di svolgere appieno il suo mandato. Lo abbiamo ribadito ieri nella sessione speciale del Consiglio di sicurezza dedicata al Libano, dove è intervenuto su mia istruzione l'ambasciatore Massari. Libano e Gaza sono strettamente legati, quindi occorre una strategia condivisa per la regione. Il cessate il fuoco a Gaza è l'elemento chiave: è questo il filo conduttore della nostra azione diplomatica nelle ultime settimane. A New York ho voluto convocare una riunione dei Ministri degli esteri del G7 e abbiamo ribadito con grande forza e unità l'invito a tutti gli attori coinvolti ad esercitare moderazione e a impegnarsi in un percorso negoziale; è quello che abbiamo fatto in occasione di tutti i G7. È indispensabile utilizzare tutti i canali di comunicazione a nostra disposizione. Sempre a New York ho incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Anche a nome del G7, ho ribadito l'urgente necessità di fare pressione su Hezbollah, sugli Houthi e sulla stessa Hamas. Abbiamo sempre deplorato le azioni destabilizzanti di Teheran, ma il canale di dialogo deve rimanere aperto. Chiediamo a tutti - assolutamente a tutti, anche a Israele - di interrompere questo drammatico ciclo di violenza e distruzione. Abbiamo anche deciso di nominare un ambasciatore in Siria proprio perché la situazione è drammatica. Ci sono rifugiati siriani che possono rientrare in quel Paese e, pur non condividendo e condannando le scelte del regime di Assad, riteniamo giusto che possa esserci un occhio italiano su questa situazione in continua evoluzione. Anche questa è stata una decisione politica. Mi spiace che chi si interessa così tanto alla politica estera si sia andato a prendere il caffè. Per evitare che tutto il Medio Oriente finisca nell'abisso di una guerra generalizzata, la via diplomatica è l'unica che può fermare una spirale di violenza e instabilità che è già durata fin troppo.

È vero che non possiamo fare quello che gli Stati Uniti da soli, la Cina da sola e la Russia da sola non riescono a fare. Sono d'accordo con lei e non lo pretendiamo. Tuttavia, l'Italia ha una tradizione diplomatica di relazioni nel Mediterraneo e con il mondo arabo, di rispetto di rispetto della cultura giudaica e di accoglienza e vicinanza alle comunità ebraiche che le può permettere di osare molto di più. È il tempo di osare per rimettere al centro più la politica, che la forza. Va detto con chiarezza a tutti: la politica e non la forza. È tempo di osare per rimettere al centro la diplomazia, più che il tema delle forniture o degli schieramenti militari. È il tempo di rimettere al centro il rafforzamento delle istituzioni internazionali. internazionali. Come è possibile che si possa dichiarare persona non gradita il Segretario generale dell'ONU? Come è possibile? L'Italia deve stare al fianco delle organizzazioni internazionali,

Non vi è stato alcun evento più drammatico di quello del 7 ottobre sul suolo di Israele dopo le guerre che conosciamo; non vi è stato alcun evento più drammatico a Gaza di quello delle morti di decine di migliaia di

E bisogna che la nostra Presidenza G7 sia usata per questo tempo straordinario, per dire a tutti che la nostra Costituzione ci impone di ripudiare la guerra come mezzo per la risoluzione dei conflitti internazionali e che (ce lo dice lo stesso articolo) siamo disponibili,

Tutti coloro che si rifanno alla civiltà occidentale rispettino quei principi e non pensino di poter imporre un ordine mondiale rispetto a un altro. Questo è il punto su cui noi dobbiamo essere molto fermi. Molto fermi. *(Brusìo).* Io non ho detto che lei lo ha detto, però lasci dire a me.

gli stabilimenti ex ILVA costituiscono asset di altissimo valore strategico per il Paese, poiché su di essi viene declinata, di fatto, la politica del Governo nel settore siderurgico. Essi compongono un complesso industriale che mette in rete 9 siti produttivi logistici e centri di servizio; in considerazione del loro profilo strategico, l'attuale Governo ha inizialmente emanato il decreto-legge n. 2 del 2023, relativo

a seguito dell'aumento dei costi energetici e porre in essere gli interventi necessari per salvaguardare la produzione, compatibilmente con gli obiettivi di tutela ambientale e di salute dei cittadini; tuttavia, la situazione gestionale e produttiva ha reso necessario ricorrere all'amministrazione straordinaria. Il 20 febbraio 2024, il controllo della società è stato trasferito a commissari nominati dal Governo. Il decreto ministeriale è stato emanato a seguito dell'istanza del 18 febbraio,

Obiettivo di questa nuova gestione commissariale era quello di rilanciare la macchina produttiva con piani di manutenzione e salvaguardia degli stabilimenti e di tutela dei lavoratori. Con le finalità della continuità produttiva sono già stati altresì varati ingenti finanziamenti, tra i quali quelli autorizzati con decreto-legge n. 63 del 2024. Ciò premesso, si chiede di conoscere lo stato dell'arte del dossier *ex* Ilva, con particolare riguardo alla presenza dei soggetti interessati all'acquisto e alle prospettive future degli stabilimenti.

abbiamo rilanciato il sito produttivo con i lavori di manutenzione necessaria, avviato il piano di ripristino degli impianti. Tra pochi giorni sarà riattivato l'altoforno 1, chiuso due anni fa. Abbiamo nel contempo attivato il pagamento dei creditori. Ripeto: in appena sette mesi già le aziende dell'indotto stanno ricevendo quanto dovuto. Le stesse aziende ancora attendono da dieci anni i crediti della precedente amministrazione straordinaria. Tutto ciò è avvenuto in un clima di piena condivisione sociale. Per la prima volta i sindacati hanno siglato l'accordo per la cassa integrazione, consapevoli che ciò avrebbe consentito la realizzazione del programma di ripristino produttivo-occupazionale. In questi pochi mesi, nel contempo, abbiamo attivato la procedura di assegnazione a nove *player* industriali. Un caso straordinario di efficienza della pubblica amministrazione nelle condizioni di maggiori difficoltà in quello che era considerato da tutti il simbolo del disastro industriale italiano. Il 20 settembre, pochi giorni fa, al termine della prima fase della procedura di vendita, sono pervenute quindici manifestazioni di interesse da parte di diversi *player* nazionali e internazionali: con riferimento all'intero complesso aziendale, dieci con riferimento a singoli rami di azienda, due con riferimento a un singolo bene. Ora inizia la seconda fase, dove coloro che hanno manifestato interesse, ma anche altri, ove volessero intervenire in questa fase, potranno ottenere le informazioni necessarie al fine di formulare poi la loro proposta complessiva. Confidiamo che la procedura possa chiudersi con l'assegnazione di tutto l'*asset* produttivo in blocco ad un unico *player*, che abbia le capacità imprenditoriale e la visione per guidare questi stabilimenti verso un futuro produttivo solido e competitivo sulla strada della tecnologia *green*. Se non si frappongono ostacoli, sempre possibili in un percorso così difficile, l'assegnazione potrebbe avvenire già agli inizi del prossimo anno, dunque ad appena un anno dal nostro intervento di commissariamento. Ci sprona, nel far bene, il desiderio di rivalsa degli operai di Taranto, di Genova di Novi Ligure e di Racconigi che io ho incontrato, visitando le fabbriche una per una, per spiegare loro qual era il percorso.

Signor Ministro, sono assolutamente soddisfatto della sua risposta, soprattutto per ciò che si è fatto per le aziende creditrici che gravitano intorno a un'importante azienda non solamente a livello nazionale, ma a livello europeo, e quindi per l'attenzione che si è dimostrata soprattutto per l'importanza che riveste quello stabilimento

secondo i dati dell'Istat leggiamo che la produzione industriale è diminuita dello 0,9 per cento su base mensile da luglio, realizzando su base annua la diciottesima frenata consecutiva. Nella media del periodo maggio-luglio si registra un calo del livello della produzione dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo tendenziale dell'anno è del 3,3 Il *trend*, signor Ministro, è preoccupante: non cresce nessun macro comparto manifatturiero, dove si registrano cali diffusi tra beni di consumi durevoli e no. L'unica eccezione è rappresentata dalle aziende dell'energia, dove si registrano incrementi tendenziali dell'1,5 Quello che emerge, signor Ministro, dagli ultimi dati è una fotografia impietosa del sistema industriale italiano. Ora, rilevato che il piano industriale di bilancio di medio termine, quello che è stato trasmesso da poco alle Camere, pone tra gli obiettivi strategici generali la definizione di una politica industriale volta a superare le disuguaglianze territoriali e le residue restrizioni alla concorrenza, e le previsioni del Piano sembrano però totalmente - e dai dati letti in precedenza sembra vero - scollegate dal quadro sopra delineato. Si legge infatti che, nel quadriennio 2026-2029, gli investimenti continueranno a fornire un deciso impulso alla crescita e, ad eccezione del 2027, ad aumentare ad un ritmo superiore a quello del PIL, anche sull'onda della spinta finale dei progetti del PNRR, inclusi gli incentivi legati al pacchetto Transizione 5.0. Ora, in merito allo stato dei progetti PNRR, signor Ministro, i ritardi accumulati dal Governo ormai sono noti a tutti e sono anche disastrosi. Ma riguardo agli incentivi del pacchetto Transizione. 5.0, proprio a causa dei ritardi del Ministro in indirizzo nell'emanazione dei provvedimenti attuativi, è ancora difficile prevedere l'impatto che dette misure avranno sulla competitività delle imprese e se davvero potranno poi contribuire in modo così incisivo alle ottimistiche previsioni di crescita, visto che solo 70 milioni sono i crediti complessivi di cui solo la metà, fino ad oggi, sono stati autorizzati. Ora, signor Ministro, io le chiedo quali iniziative intenda concretamente porre in essere per contrastare l'attuale calo della produzione industriale e per raggiungere gli obiettivi di crescita delineati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine che, alla luce dei dati e delle considerazioni espresse in premessa, appaiono irrealistici. inoltre se non ritenga invece opportuno rimediare ai ritardi accumulati nell'attuazione delle misure legate agli incentivi del piano Transizione 5.0, prevedendo prioritariamente una proroga in favore delle imprese per la messa in funzione degli investimenti e convocando un tavolo con le associazioni di categoria

il quadro reale e complessivo della situazione. L'Italia reagisce meglio degli altri grandi Paesi industriali europei, molto meglio di Germania e Francia. In un mondo in cui le guerre sono intorno all'Europa e si spezzano le catene di approvvigionamento, si chiudono i mercati e il nostro più grande *partner* industriale entra in recessione, il nostro Paese segnerà quest'anno una crescita del PIL dell'1 per cento, più della media europea, avendo anche nel contempo il più basso tasso di inflazione d'Europa. Supereremo il Giappone come quarto Paese esportatore al mondo e continueremo ad aumentare l'occupazione; in dodici mesi sono stati creati altri 496.000 posti con contratti stabili, che segnano il *record* storico di occupazione in Italia. Il tasso di disoccupazione è infatti sceso al 6,2 Dopo il taglio del reddito di cittadinanza, è questo il momento del riscatto del lavoro italiano. Il Piano strutturale di bilancio rappresenta un passo importante per l'industria italiana, investe sulle imprese e non lascia indietro nessuno. Anche per questo abbiamo realizzato il piano Transizione 5.0, che si affianca, si somma e non sostituisce Industria 4.0. E' l'unico piano europeo che coniuga le due transizioni, mettendo a disposizione delle imprese in questo biennio quasi 13 miliardi di euro. Esso, inoltre, a differenza dei piani precedenti, è finanziato con risorse europee e per questo ha regole che abbiamo dovuto concordare con la Commissione. Sono che abbiamo ricavato dalla revisione, contrastata dal suo partito, dei programmi del PNRR, che è stata realizzata dopo il necessario passaggio parlamentare nel dicembre dello scorso anno. Proprio per questo, essendo risorse del REPowerEU, non è possibile prevedere una proroga delle misure e non è possibile apportare modifiche sostanziali senza nuovi e defatiganti confronti in sede europea che impiegherebbero altri mesi, rendendo impossibile l'uso delle risorse da parte delle imprese nei tempi cogenti del PNRR. Infine, per quanto riguarda il dialogo con le associazioni di categoria, posso assicurarle che ciò avviene ed è continuativo, cosa che invece spesso è mancata in passato per analoghe misure automatiche, come ben sanno le imprese che hanno utilizzato il credito ricerca e sviluppo e a cui noi abbiamo intenzione di porre rimedio nella prossima manovra economica. Il piano Transizione 5.0 è il piano più avanzato in Europa, l'unico che coniuga le due transizioni digitale e *green* e l'unico che consente anche la formazione dei lavoratori (fino al 10 per cento delle risorse è possibile destinarlo anche alla formazione dei lavoratori). Per questo riteniamo che sia strategico nella strada verso un'industria più competitiva, sostenibile e sicuramente ancor più capace di conquistare gli spazi di mercato che i dati dimostrano il *made in Italy* può fare. mi rivolgo a lei tramite il Presidente. I dati forniti sono quelli che leggiamo dal «Sole 24 Ore», tra l'altro riportati non solo da noi: crolla la domanda di *robot*, quindi di macchine utensili, del 26 per cento e, tra l'altro, il presidente Rosa dell'Unione delle aziende produttrici di macchine utensili dice che la colpa è

Come può arrivare a questo numero, se poi entro dicembre 2025 la misura scade e non c'è un piano di previsione almeno triennale? È quello che prevedeva anche Transizione 4.0 e non è vero che lei è andato in continuità, perché quel piano l'ha soppresso. Non è vero che sono cumulabili: sono misure assolutamente non cumulabili. Interrotta la

Non c'è crescita. caso amaro della produzione industriale italiana - il Governo Conte II aveva mancato di opporre la *golden power,* quando ricordo che al parlamentare Urso, durante un'interrogazione fatta all'allora ministro dello

dagli ultimi dati disponibili, i grandi gruppi del mercato del lusso, come Lvmh e Kering, hanno fatto registrare per il 2024 un importante calo degli ordini presso i fornitori italiani. Il nostro Paese è caratterizzato dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell'alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*. L'industria italiana di alta gamma vale 144 miliardi di euro e fornisce un contributo al PIL del 7,4 per cento, con una quota dell'*export* di circa il 50 Il settore coinvolge quasi 2 milioni di occupati diretti e indiretti e rappresenta una delle tante eccellenze nel mondo dell'Italia, che racchiude la nostra storia, la nostra cultura e le tradizioni del nostro Paese. Ogni Regione si distingue, infatti, per le sue specificità, le quali, mescolandosi con la creatività e l'abilità del lavoro degli artigiani, riescono ad esaltare quell'unicità e la diversità dei nostri territori. Il saper fare è l'elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività. Tale patrimonio, però, rischia di essere disperso nel corso dei prossimi anni per via delle difficoltà in cui versa il settore dell'alta gamma. Il problema principale della carenza dei giovani che intendono investire nel settore dell'alta gamma, perché è divenuto negli anni sempre meno attrattivo, rappresenta il più grande ostacolo allo sviluppo competitivo competitivo dell'artigianato di alta gamma. A questo, poi, si aggiungono altre criticità che vanno dalla stentata digitalizzazione alla micro e piccola dimensione delle imprese, che rende spesso difficile la loro internazionalizzazione. L'Unione europea ha recentemente approvato il regolamento 2411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Esso modifica i regolamenti precedenti e va ad istituire un sistema di produzione delle indicazioni geografiche per i prodotti di eccellenza. Ciò premesso, le chiedo, signor Ministro, quali azioni immediate intenda intraprendere per rilanciare e promuovere la crescita e lo sviluppo del settore

la tutela e il rilancio del *made in Italy* è il fulcro dell'azione del Governo, come dimostra anche la nuova denominazione dello stesso Ministero, che identifica una chiara *mission* di politica industriale. In tal senso, la legge quadro sul *made in Italy* approvata dal Parlamento contiene una serie di disposizioni a tutela del sistema industriale italiano, con un *focus* particolare proprio sui settori dell'alta gamma. Abbiamo introdotto, appunto, l'indicazione geografica per prodotti artigianali e industriali nel nostro ordinamento. Il relativo bando è attivo fino al 31 ottobre per l'erogazione di un contributo per supportare le imprese nella predisposizione del disciplinare di produzione di prodotti industriali e artigianali tipici in sede europea. Sempre nel citato disegno di legge quadro sul *made in Italy*, abbiamo realizzato ulteriori misure per la promozione della formazione professionale, la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e l'internazionalizzazione delle aziende. Abbiamo istituito la Giornata nazionale del *made in Italy* anche per ispirare le nuove generazioni; il Premio per il maestro del *made in Italy* per i settori dell'alta gamma (tessile, arredamento, cantieristica e agroindustria), e il Liceo del *made in Italy*, già aperto in tempi *record* con i primi 30 corsi in quasi tutte le Regioni italiane. In tema di digitalizzazione, ricordo il Piano transizione 5.0, che vede 13 miliardi di euro nei prossimi due anni in crediti fiscali, per la prima volta, a differenza dei precedenti piani, utilizzabili appieno proprio dalle piccole e medie imprese, anche per la formazione del loro personale. Altre misure incentivanti per le piccole e medie imprese sono ovviamente reperibili nel portale del Ministero. del Ministero. Ad esse è dedicato anche il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che solo lo scorso anno ha garantito finanziamenti per circa 46,2 miliardi di euro, rispondendo alle esigenze di liquidità in questa difficile fase congiunturale. Inoltre tra poche settimane vedrà la luce la prima legge annuale per le piccole e medie imprese, prevista in un dispositivo di legge del 2011 e mai realizzata dai Governi nei tredici anni precedenti. Si tratta di una legge annuale sulle piccole e medie imprese e sull'artigianato che anno dopo anno, a cominciare da quest'anno, tenderà a semplificare, incentivare e sostenere le attività delle piccole e medie imprese. Noi siamo pienamente consapevoli che le PMI sono la forza del nostro sistema e faremo di tutto per rafforzarne la loro eccellenza.

nel mondo hanno senso solo se la terza è *Italy*. Può sembrare banale, ma *made in* *France*, in *Nederland* o in *Belgium*, non hanno quel valore aggiunto. *Made in Italy* è uno dei primi dieci *brand* al mondo e, nonostante tutto, per una situazione congiunturale, tante aziende stentano ad arrivare alla fine del mese. Come generazione abbiamo sbagliato una cosa. Noi abbiamo detto ai nostri figli "se non studi, vai a lavorare": avremmo dovuto dire "se studi, vai a lavorare". Facendo questo, abbiamo allontanato i nostri figli da quel lavoro fatto

Firenze. Sicuramente l'IGT è una grande opportunità e tutte le misure che la Lega, questo Governo e lei, signor Ministro, stiamo mettendo in atto tutti insieme credo possa essere un'importante sfida, una grande opportunità per far tornare ai nostri figli l'orgoglio di fare quel lavoro con le mani che ha fatto tanto grande questo Paese.

il settore dello spazio sta attraversando in questi anni una nuova fase di sviluppo, diventando un campo di confronto sempre più rilevante per le economie nazionali. Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge in materia di economia dello spazio che, una volta approvato dal Parlamento, costituirà la prima legge quadro in materia spaziale nel nostro ordinamento, ponendo l'Italia all'avanguardia nel mondo e anticipando le intenzioni dell'Unione europea in merito a un regolamento per il settore. L'Italia è protagonista della nuova era con i suoi astronauti e con le sue imprese e ha un peso sempre maggiore nell'European Space Agency, con il sesto posto al mondo per investimenti nel settore in proporzione al PIL con 4,6 miliardi di euro allocati solo nel 2023, potendo contare su un comparto industriale che vede attive 250 imprese, 15 distretti e 6.000 addetti. In un'intervista i sindaci rispettivamente di Cannes e di Tolosa - due città molto competitive nel settore dell'aerospazio hanno dichiarato che si è dinanzi ad un sorpasso dell'Italia rispetto alla Francia per la crescita del settore aerospaziale. Dal 14 al 18 ottobre, Milano ospiterà la 75ª edizione dell'International astronautical congress. La città lombarda è stata selezionata dagli oltre 400 delegati dell'assemblea generale dell'International Astronautical Federation, anche in virtù degli investimenti previsti dal Governo nel settore spaziale, che testimoniano l'impegno dell'Italia a diventare *leader* in questo campo. Si prevede la partecipazione di migliaia di esperti del mondo dell'industria, della ricerca e delle istituzioni, espressione del fiorente ecosistema globale di *start up*, imprenditori, laboratori, ricercatori e produttori coinvolti in attività spaziali. L'edizione di quest'anno svilupperà i temi legati a un uso più consapevole e responsabile dell'ambiente spaziale, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale, evidenziando l'importanza di mantenerlo sicuro e aperto all'esplorazione, all'uso pacifico e alla cooperazione internazionale da parte delle generazioni presenti e future, nell'interesse del pianeta e di tutte le Nazioni. Si chiede di sapere quali siano gli obiettivi che il Governo intende perseguire con la sua politica aerospaziale e quali misure intenda adottare per garantire che l'Italia raggiunga i più alti livelli nel settore.

anche per questo abbiamo realizzato la prima legge italiana sullo spazio, che ora è sottoposta all'esame del Parlamento; una legge che colma un vuoto nell'ordinamento, regolando l'accesso allo spazio anche per gli operatori privati - perché oggi nello spazio vanno soprattutto i privati - supportando le piccole e medie imprese e le *start up* del settore e incentivando investimenti a lungo termine. In tal modo il nostro Paese si pone all'avanguardia in Europa, in attesa del regolamento europeo annunciato, ma ancora non realizzato. Lei ha citato l'importantissimo *meeting* del Congresso internazionale astronautico, che si terrà nei prossimi giorni a Milano con decine di migliaia di partecipanti, che testimonia quanto significativo sia diventato il ruolo dell'Italia in questa economia del futuro. L'Italia è al sesto posto per investimenti. Lei ha citato quanti miliardi sono stati allocati nel 2023; da qui al 2026 abbiamo già allocato 7,3 miliardi di euro, includendo fondi nazionali, europei e fondi del PNRR. Questi fondi ci permettono di sviluppare un ecosistema fatto di grandi imprese, ma anche di tante piccole e medie imprese, in 15 distretti, quindi in quasi tutte le Regioni d'Italia. Diversi progetti dimostrano il senso della nostra strategia. Ricordo Earth Moon Mars, volto a creare una rete di collegamenti tra Terra, Luna e Marte, e il progetto ORACLE, che mira a estrarre ossigeno dalla regolite lunare, rendendo così possibile la permanenza prolungata di esseri umani sulla Luna (progetti italiani). Abbiamo anche rafforzato da subito la cooperazione internazionale con Francia e Germania, siglando un'intesa per l'autonomia europea nel settore dei lanciatori, con particolare attenzione a Vega C e Ariane 6. Quest'accordo, promosso dall'Italia con gli altri grandi attori spaziali europei, garantirà un accesso europeo indipendente allo spazio, cruciale per la sicurezza e la competitività globale. Nel settore delle telecomunicazioni spaziali, il Centro spaziale del Fucino è stato scelto come centro di controllo per il sistema europeo IRIS2, con il raddoppio della base italiana. In Sicilia sarà realizzato l'osservatorio dell'ESA per individuare i più lontani corpi celesti e prevenire da eventuali ricadute. Senza il nostro intervento e la nostra assunzione di responsabilità, rischiava di venire spostato nelle Canarie. Ora, forti di questo, supportiamo la candidatura del sito in Sardegna per la costruzione del grande Telescopio Einstein. Infine, e su tutti, ricordo dove è nata l'avventura spaziale dell'Italia, l'Africa. Sono tornato poche ore fa dalla mia missione in Kenya, dove ho visitato il Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi. Lì nascerà il centro di formazione per lo sviluppo della politica spaziale dei Paesi africani: un centro di formazione, un centro di avvistamento e di rilevazione e in futuro anche un centro per il lancio di satelliti di piccola dimensione, proprio per i programmi dei Paesi africani, nelle piccole costellazioni dei loro Paesi. Anche questo fa parte del Piano Mattei, di una logica che vuole fare dell'Africa un *partner* tecnologico, scientifico e industriale di grande rilevanza; una logica in cui l'Italia può svolgere un ruolo determinante, come loro stessi ci riconoscono.

della giurisdizione dell'economia dello spazio. Era un *vulnus* da colmare e questo è stato fatto con un atto che oggi spetta a noi del Parlamento portare a termine e magari perfezionare, con il contributo di tutte le forze politiche, perché siamo di fronte a passi importanti che l'Italia sta compiendo nel panorama internazionale, sfidando in maniera avveniristica la storia.

negli equilibri internazionali - se vogliamo, il mondo e l'industria spaziale contribuisce, da questo punto di vista - su un *asset* specifico che è avveniristico per definizione; è un *asset* che può cambiare il mondo in termini prospettici. È un po' la nuova industria del futuro e l'Italia è appieno parte integrante di questo percorso; pertanto non è più soltanto *leader* storico della componentistica, come da sempre il nostro *know-how* ci consente di vantare, ma oggi esploriamo mondi nuovi; andiamo con il Piano Mattei in Africa,

nel Fucino, ad Avezzano, quando abbiamo conosciuto da vicino Iris2, con tutto quello che di avveniristico ci sarà da qui ai prossimi anni. Per questo e non soltanto per questo, per quello che so essere una sua passione nell'ambito dell'economia spaziale e dell'industria aerospaziale, ringraziandola per la cura